in merito alle interrogazioni, il Ministero dello sviluppo economico precisa che, pur non essendo stato qui coinvolto nella questione illustrata dall'atto di sindacato, segue gli sviluppi della situazione del centro di ricerche Nerviano Medical Sciences nell'ambito delle attività del tavolo permanente per il settore farmaceutico istituito presso lo stesso Ministero. La vertenza infatti è seguita presso la Regione Lombardia. Dalle informazioni assunte dal Ministero presso la medesima Regione risulta che, nel maggio 2009, è stato ultimato l'*iter* di ricapitalizzazione della Nerviano Medical Sciences (NMS) srl. Ciò è avvenuto mediante la cessione del credito, di 30 milioni di euro, di Unicredit verso NMS alla proprietà, Congregazione dei figli dell'Immacolata concezione. Quest'ultima a sua volta ha provveduto a ricapitalizzare NMS per lo stesso importo. La Regione Lombardia sta portando avanti gli impegni presi a favore della Nerviano Medical Sciences a seguito della suddetta ricapitalizzazione e sta promuovendo un percorso finalizzato allo sviluppo strategico del centro di ricerca. In particolare, sono ancora in corso altri incontri presso la Regione, sia per la maggior definizione del piano industriale, che è stato presentato in data 10 novembre 2009 dalla società, sia per trovare soluzioni al fine di rendere concreto il rilancio del centro di ricerca. Le organizzazioni sindacali hanno valutato positivamente il valore strategico del piano di sviluppo presentato, poiché contiene i presupposti, alcuni dei quali dovranno essere consolidati, per un rilancio competitivo sul mercato del centro stesso. Tra i punti qualificanti del piano è prevista la nascita di un centro universitario (NMS Accademia), che potrebbe garantire una *partnership* stabile con la Regione favorendo l'occupazione. Comunica, inoltre, la Regione che i prossimi passaggi sono, quindi, relativi, da un lato, al proseguimento della trattativa con Pfizer, che sta procedendo nei tempi programmati, e, dall'altro, all'attivazione di nuove *partnership*. Risulta, ancora, che il centro, proprio al fine di favorire, accanto agli aspetti scientifici e di *business*, anche l'ambito finanziario fortemente connesso ai programmi di rilancio del centro ricerche, ha recentemente rinnovato i propri organi sociali. La Regione, ha informato infine, per le vie brevi, circa la possibilità di un proprio finanziamento triennale, attraverso l'assessorato alla sanità, al centro medesimo per la ricerca oncologica. Il Ministero del lavoro comunica, infine, che allo stato attuale non risulta pervenuta alcuna domanda di cassa integrazione relativa al Nerviano Medical Sciences. Il Ministero dello sviluppo economico è totalmente a disposizione per ogni supporto possa essere necessario per la migliore definizione degli interventi del nuovo piano industriale, così come a convocare un tavolo di confronto con tutte le parti interessate, qualora fosse richiesto.

del presidente della Commissione bilancio Fabrizio Cecchetti, ha attivato un finanziamento di 15 milioni di euro (che è sicuramente una misura importante), ma è anche vero che la ricerca è un bene nazionale. Quindi, se anche da parte dello Stato, in caso di necessità,

per effetto della grave crisi finanziaria, ha rischiato il fallimento. Poi vi sono stati gli interventi che il Vice Ministro correttamente ricordava e, fortunatamente, si è riusciti ad impedirlo. Tuttavia - ed è l'altra ragione per la quale non mi ritengo

non è stato rinegoziato l'accordo con Pfizer, il che sta determinando un livello di costi assolutamente insostenibile, per cui c'è il rischio che, se non nel 2010, nel 2011, per effetto

cui abbiamo l'ennesimo caso in cui si chiedono intervenenti giusti di ricapitalizzazione alle banche, con il contributo degli enti locali, e poi la proprietà non mette non mette una lira. Così come - e concludo - è del tutto evidente che rimane a rischio il futuro del centro di ricerca farmacologica di Nerviano che, voglio ricordarlo anche in quest'occasione, occupa 800 dipendenti, di cui 650 ricercatori.

per sollecitare interventi sul piano finanziario, sia per trovare nuovi partner industriali, perché solamente con un intervento che abbia questa duplice caratteristica si possono creare le condizioni per determinare un futuro migliore al centro di ricerca di Nerviano.

un articolo di Massimo Numa dal titolo «Una molecola killer ha ucciso 27 eroinomani - La scoperta dopo gli esami della Scientifica». In questo articolo si riportava la notizia che i laboratori della Polizia scientifica avevano individuato uno stupefacente oppioide particolare, denominato «6-Mam», di provenienza afgana, che avrebbe provocato la morte di questi 27 cittadini tossicodipendenti, in Provincia di Torino, nell'estate del 2009. L'articolo riportava anche le dichiarazioni del professor Giovanni Serpelloni, direttore del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, che cito: «Alcuni cadaveri sono stati trovati con ancora le siringhe conficcate nelle braccia. Una morte fulminea. Il tempo di assimilazione della molecola è di pochi secondi, molto più veloce dell'eroina (...). Allora, non fu perso un solo istante. Decidemmo di istituire il livello di massima allerta 24 ore dopo avere ricevuto, dagli organismi locali, i dati sul numero e sulle circostanze dei decessi. Ma il caso Torino è stato unico in Italia, in quel periodo, e ci ha consentito di studiare a fondo ogni dettaglio di questa vera e propria strage». Rispetto al perché era stato immesso sul mercato criminale uno stupefacente così letale, Serpelloni dichiarava: «Impossibile ricostruire questo tipo di scenari, noi possiamo solo accertare il tipo di sostanza utilizzata, le caratteristiche chimiche, le aree di provenienza. E cercare di evitare, in futuro, con la prevenzione, una catena di morti di queste dimensioni spaventose»; considerato che il decreto 23 gennaio 2009 del Sottosegretario di Stato alle Politiche per la Famiglia, per il Contrasto alle Tossicodipendenze e Servizio Civile le politiche antidroga), così recita: «Il Dipartimento, mediante sistemi di allerta precoce e il coordinamento delle altre amministrazioni centrali coinvolte, provvede alla sorveglianza epidemiologica, delle caratteristiche delle sostanze stupefacenti circolanti, dei comportamenti di abuso e dei fenomeni droga correlati, per l'evidenziazione precoce dei rischi e delle possibili conseguenze rilevanti per la salute della popolazione»,

ha dato ulteriori informazioni, spiegando: «La segnalazione di un numero particolarmente elevato di overdose infauste nell'area torinese da parte di un'associazione di volontariato operante nella Regione Piemonte

una complessa indagine di campo per poter avere una risposta interpretativa del fenomeno che fosse esauriente al fine di lanciare un'allerta soprattutto diretta ai consumatori». Dopo due mesi, un'allerta immediata è davvero difficile. «Come è stato successivamente evidenziato dai dati raccolti, dopo aver lanciato l'allerta il numero delle overdose è drasticamente crollato». Ormai erano già praticamente morti tutti, perché l'evento risaliva a due mesi prima. «Quindi è stato proprio grazie all'allerta che i consumatori sono stati avvisati del grave pericolo evitando ulteriori morti. Dopo l'attivazione dell'allerta la collaborazione con le strutture regionali, la magistratura, le forze dell'ordine e le strutture sanitarie coinvolte è stata particolarmente efficace e ben organizzata. Il ritardo nell'attivazione dell'allerta non può essere imputato al Sistema nazionale ma, in caso, ad una scarsa sensibilità informativa dei sistemi e degli osservatori locali, oltre che ad una oggettiva difficoltà da parte delle unità di primo rilevamento di percepire il fenomeno nelle sue fasi iniziali. Ciò, eventualmente, denota la necessità di attivare forme di collaborazione sempre più intense tra strutture locali (che dovrebbero essere in grado di percepire più precocemente i primi segni ed eventi negativi trasformandoli in vere e proprie segnalazioni) e il Sistema nazionale, che è in grado d'intervenire a più ampio raggio e molto più tempestivamente, attivando allerte che possono interessare altre Regioni quando non addirittura l'intero territorio nazionale». Serpelloni domanda da porsi, al fine di migliorare i sistemi, dovrebbe essere quindi quella del perché non hanno funzionato i sistemi locali e perché il Sistema di allerta nazionale non sia stato avvisato più precocemente, considerate la capacità, la tempestività e gli accessi che il Sistema possiede e che avrebbero potuto determinare un'azione più immediata da parte di tutti gli enti e le strutture locali coinvolte». Non credo sia opportuno in questa situazione fare lo scaricabarile, a ciascuno il suo e, in particolar modo,

morti per *overdose* citate in premessa; tenendo conto che solamente una piccola parte dell'opinione pubblica (i lettori dell'articolo de «La Stampa» citato in premessa) è venuta a conoscenza dei risultati dei laboratori della Polizia Scientifica non durante l'*escalation* delle morti

se non reputi che la presenza di una o più narcosale nella città di Torino - sull'esempio di quelle operanti da un ventennio in varie città europee - avrebbe evitato alcune di quelle overdose. Del resto, la riduzione del danno è uno dei quattro pilastri delle politiche europee di contrasto alla tossicodipendenza. se non pensi che l'utilizzo dell'oppio afgano per produrre morfina - come proposto prima dai radicali poi dal Parlamento europeo - avrebbe impedito la trasformazione di quell'oppio in eroina e, nel caso specifico in «6-Mam», il conseguente smercio sulla piazza criminale torinese e la conseguente morte di 27 27 persone, e se, alla luce delle considerazioni esposte, non ritenga che il regime proibizionista esistente su alcune droghe sia il vero responsabile dei 27 decessi per overdose a Torino nell'estate del 2009

per determinate materie, mentre sono rimaste al Governo nazionale solo le competenze residue di coordinamento e programmazione. Ricordo solo un dato, perché mi compete: l'intero Dipartimento, a livello nazionale, ha 9 milioni di euro per tutte le attività che deve svolgere, mentre giorni fa ho seguito con interesse la presentazione del programma della Regione Piemonte, che stanzia 60 milioni di euro per le tossicodipendenze. E non è che il Piemonte sia un'eccezione: è che l'intero fondo che una volta era in capo allo Stato è stato trasferito alle Regioni, insieme alle competenze che, per esempio, riguardano l'organizzazione dei servizi (SERT), che non sono più dello Stato, ma delle Regioni. È quindi con un certo imbarazzo che devo dire che,

del verificarsi degli eventi, ma non aveva fatto pervenire alcuna segnalazione al livello nazionale. Ebbene, nessuno ha la scienza infusa: se sul territorio chi ha la competenza non segnala e la segnalazione poi arriva da altre parti, nessuno può essere in grado di sapere quello che accade in Sicilia o in Calabria, piuttosto che in Piemonte. Tuttavia, non appena è arrivata questa unica segnalazione da parte di un'associazione di volontariato piemontese, in

scoperto che la mortalità dei casi segnalati era dovuta all'assunzione di un particolare tipo di eroina, denominata *Black Tar* a causa del suo particolare colore, che era disponibile sulle piazze di spaccio dell'area piemontese, in tale sostanza era presente un'elevata percentuale di una molecola monoacetilmorfina, causa dei decessi. decessi. Confermata la pericolosità, alle ore 12,36 del 14 luglio, il Sistema attivava il massimo grado di allerta e non solo in Piemonte, ma avvertendo tutte le Regioni italiane, i laboratori, le forze dell'ordine e anche

Il 15 settembre 2009, dopo 40 giorni dalla registrazione dell'ultimo caso, come da protocollo standard, e soprattutto in considerazione del fatto che non veniva riscontrata un'ulteriore presenza sul mercato clandestino della sostanza, il Dipartimento antidroga, sempre attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce, inviava una nuova informativa in cui si comunicava la chiusura dell'allerta. A conclusione delle procedure di analisi della dinamica dei decessi, i tecnici del Dipartimento antidroga, in sede di consuntivo delle operazioni, hanno potuto rilevare carenze nell'attività di segnalazione dei decessi da parte delle quando si parla di collaborazione, è evidente che un sistema funziona se i terminali locali, quando succede qualcosa, comunicano tempestivamente quello che sta accadendo. Inoltre, visto che siamo in un sistema ormai federale regionale e vi sono 20 Regioni con le quali fare i conti, ogni Regione ha proprie procedure e modalità di approccio al fenomeno della droga. droga. La segnalazione è arrivata in ritardo, ma è anche vero che dopo l'allerta il fenomeno è rapidamente scemato e non

attivarsi per impedire nuovi decessi. Sicuramente, e questo è un problema di cui abbiamo lungamente parlato a Trieste, durante la Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze, è assolutamente necessaria una più stretta collaborazione

per il recupero dei tossicodipendenti, rispetto ad altre che stanziano pochissimo. D'altronde, è totalmente discrezionale da parte delle Regioni utilizzare o non utilizzare una parte del Fondo sanitario in direzione del recupero dei tossicodipendenti. È altrettanto vero che la Costituzione attuale impedisce

sia destinato, come accadeva una volta con il fondo nazionale, al campo della prevenzione e del recupero dei tossicodipendenti. Ricordo anche - recentemente ne ha parlato qualche trasmissione televisiva

e purtroppo questo succede spesso a ragazzi giovanissimi, che muoiono per l'assunzione disinvolta di tali sostanze. Proprio attraverso il monitoraggio di quei ricoveri ospedalieri, siamo stati in grado, in tempo reale, da un lato, di chiedere l'inserimento in tabella di queste sostanze, che contengono cannabinoidi, per cui devono essere monitorate e se ne deve rendere penalmente perseguibile lo spaccio, dall'altro, di ottenere un'ordinanza da parte del

questa posizione è stata sposata sostanzialmente da tutti gli Stati del mondo, salvo due o tre in Europa, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Giappone all'Afghanistan, dall'Australia al Canada. Tale posizione è patrimonio diffuso, tant'è vero che il documento finale è stato approvato sostanzialmente all'unanimità. Quindi, noi riconosciamo talune misure di prevenzione secondaria delle patologie correlate alla tossicodipendenza (l'epatite, le morti di droga correlate, l'infezione da HIV). Tali interventi però devono essere in maniera indispensabile e irrinunciabile mirati, da un lato, a prevenire e ridurre i rischi e i danni per la salute delle persone tossicodipendenti, derivanti da comportamenti caratteristici delle tossicodipendenze, e dall'altro a ridurre le condizioni sociali devianti di discriminazione e stigmatizzazione o il rischio di criminalità, atteso che la finalità essenziale di ogni iniziativa è un intervento globale sulla persona, che preveda il completo recupero e non la sua cronicizzazione in condizioni eticamente inaccettabili. In altri termini, tali azioni di prevenzione delle patologie correlate devono essere sempre considerate integrative e non sostitutive dell'intervento terapeutico e riabilitativo e tese a recuperare totalmente la persona, affrancarla dall'uso di qualsiasi sostanza stupefacente e reinserirla nella società e nel mondo del lavoro. Abbiamo un progetto mirato proprio a questa fase molto delicata, che è quella dell'uscita dalle comunità o dal SERT: chi esce dal tunnel della droga, naturalmente, ha bisogno di essere reinserito, trovando un lavoro e condizioni di vita normali. La distribuzione controllata di eroina si tradurrebbe nella consegna e assunzione di un prodotto farmaceutico del tutto simile alla sostanza stupefacente presso strutture dedicate a cui il tossicodipendente avrebbe accesso tre o quattro volte al giorno per praticarsi l'iniezione endovenosa. Il Dipartimento antidroga rileva, oltre alle problematiche di carattere giuridico, non può essere considerata una priorità, attesa la bassissima percentuale di soggetti che ne potrebbero usufruire (non superiore al 3 per cento della popolazione tossicodipendente). Tra l'altro, le esperienze di altri Paesi (e anche di questo si è discusso a lungo a Trieste e a Vienna), in cui la prescrizione di eroina è stata adottata, hanno mostrato che gli stessi pazienti tendono, nell'arco di quattro-sei mesi, ad abbandonare questo tipo di soluzione. Non va, da ultimo, sottovalutato l'alto costo del dispositivo sanitario necessario a supportare quest'iniziativa, con possibili ripercussioni sullo svolgimento a favore degli stessi tossicodipendenti di attività sanitarie di ben altra efficacia.

delle cosiddette narcosale, faccio presente che tale iniziativa non è supportata in Italia da alcuna previsione normativa che ne consenta l'attivazione. Tale azione, oltre che impercorribile sotto il profilo giuridico, è totalmente in contrasto con le politiche per contenere il fenomeno della tossicodipendenza adottate dal Governo sulla base delle quali si considera prioritario privilegiare l'impiego delle risorse in direzioni diverse, con l'individuazione di attività di primo contatto mediante unità mobili, *drop-in center*, centri di pronta accoglienza e offerta di terapie farmacologiche a bassa soglia. Più in particolare, è auspicata (e in molte Regioni è già stata intrapresa) l'attivazione di accoglienze immediate e l'utilizzo di terapie farmacologiche come forma di incentivazione al contatto e al proseguimento di percorsi terapeutici e di affrancamento dall'uso di sostanze stupefacenti a più alta soglia e nel più lungo termine. Come ricordavo prima, questa impostazione "italiana" - che non è ideologica, è molto pragmatica - trova importanti sostenitori anche in ambito internazionale. Non a caso, nel suo rapporto 2009, presentato nel marzo scorso, a Vienna, nel corso dei lavori della 53a della 53a Sessione della CND, l'*International Narcotics Control Board* (INBC) delle Nazioni Unite, con la formale raccomandazione n. 32, ha richiamato i Governi che hanno allestito le cosiddette "camere per l'iniezione di droghe" a "chiudere per l'iniezione di droghe" a "chiudere queste facilitazioni e soluzioni similari e a promuovere l'accesso dei consumatori di droga ai servizi sanitari e sociali, compresi i servizi per il trattamento dell'abuso di droga, in conformità con le disposizioni dei trattati internazionali di controllo sulla droga". Attualmente, la maggior parte dei sistemi regionali sono in grado - se ben orientati - di creare efficaci condizioni di primo contatto e incentivazione all'entrata in trattamento (obiettivo primario), mentre l'apertura di tali "camere del buco" potrebbe comportare lo spostamento dell'attenzione e degli impieghi di risorse verso soluzioni meno impegnative che, invece di essere aggiuntive, potrebbero correre un forte rischio di diventare sostitutive, creando così sacche di pazienti solo controllati ma non gestiti correttamente da un punto di vista terapeutico e, soprattutto, riabilitativo. Anche in questo caso le contrapposizioni ideologiche del passato sono state ampiamente superate quando una dizione equivoca come "riduzione del danno" è stata tradotta sia a livello di riduzione del rischio che di accettazione di tutte quelle terapie che possono essere adottate da alcune comunità che non fanno uso di metadone quindi sono assolutamente contrarie a terapie farmacologiche, da altre che fanno uso del metadone, da unità di strada che tentano di agganciare il tossicodipendente attraverso il suo avvicinamento ai servizi.

dalla possibilità di recupero integrale della persona tossicodipendente. Quindi, tutti gli strumenti sono validi se finalizzati a quell'obiettivo. Per quel che riguarda la possibilità

e sotto stretto controllo delle autorità locali ed internazionali, in diversi Paesi (come, ad esempio, in India). Rispetto alla domanda globale di medicinali antidolorifici, esiste attualmente un'enorme eccedenza di produzione, ben superiore alle quantità di oppio che vengono comunque immagazzinate per garantire la copertura del fabbisogno mondiale per un intero biennio. Aumentare in maniera esponenziale la richiesta per uso medico di questi medicinali, a livello mondiale, richiederebbe anni di formazione, modifiche negli ordinamenti giuridici e cambiamenti di mentalità nell'opinione pubblica che, invece, postulano tempo e grandi investimenti. Ma anche in presenza di un repentino e consistente innalzamento della domanda, l'enorme quantità di oppio prodotta in Afghanistan risulterebbe comunque esorbitante rispetto alle accennate necessità terapeutiche. luogo, la "diversione" di quote ingenti di prodotto per uso medico verso i circuiti clandestini per la sintesi dell'eroina, se è purtroppo un rischio ineliminabile anche nei Paesi dotati di sistemi normativi, giudiziari e di polizia in grado di disciplinare con regole stringenti la produzione dell'oppio, potrebbe diventare un fenomeno incontrollabile in un contesto, come quello afgano, in cui in molte zone del Paese non esiste ancora un controllo effettivo del territorio. Ne sanno qualcosa gli iraniani,

luogo, il prezzo pagato dalle aziende farmaceutiche non potrebbe in alcun modo competere con quello pagato dalle agguerrite organizzazioni criminali dedite al narcotraffico e alla produzione illecita di eroina. Ne conseguirebbe un'inevitabile involuzione dell'attività di coltivazione, solo apparentemente destinata a scopi medici, ma di fatto funzionale al mercato clandestino delle organizzazioni criminali. Da ultimo, le tecniche di coltivazione in un Paese lacerato dai conflitti armati e privo di alcun sistema di valutazione e controllo, men che meno sulla qualità dei prodotti, porterebbero alla produzione di raccolti d'oppio caratterizzati dalla presenza massiccia di impurità, tossine generate dagli antiparassitari o dagli agenti fertilizzanti, tali da renderli inutilizzabili per il successivo impiego farmaceutico e non concorrenziali rispetto a quelli ottenuti in altri Paesi con modalità e procedure ben consolidate. Quanto, infine, al cosiddetto "regime proibizionista", ricordo per l'ennesima volta che l'Italia è forse il Paese meno proibizionista del mondo. Non manco mai di ricordare ai giovani, specialmente nelle scuole, che se si recano in Cina e vengono colti con un grammo di hashish rischiano la pena capitale;

Mi augurerei comunque di non sentir più parlare nel 2010 di «tunnel della droga», perché credo davvero siano dei termini superati, così come «tossicodipendenti zombie». Credo si possa andare avanti, soprattutto se non si vuole avere un atteggiamento

anche il metadone. E allora, mi chiedo: perché l'eroina no? L'eroina comunque verrebbe fornita, lei ha detto, come un farmaco. Certo, come un farmaco, e sarebbe davvero molto diversa da quella droga e da quelle sostanze che invece circolano per strada. Lei ha poi detto che comunque nei Paesi dove sono state fatte esperienze di questo tipo in realtà

perché si assume dell'eroina ma perché quella sostanza è stata tagliata male o ha delle molecole tali che poi comportano la morte.

affermazione è molto generica, perché poi bisognerebbe cercare di capire che direzione prendono queste persone: abbandonano quel tipo di trattamento per fare che cosa? Per tornare sulla strada, oppure perché si indirizzano verso altre

sicuramente anche la domanda legale, e non quella reale, che oggi viene coperta. Lei dice inoltre che la concorrenza con il narcotraffico è proprio il proibizionismo che fa lievitare a dismisura il prezzo di una sostanza che, in realtà, è naturale. è naturale. Non ho assolutamente più tempo per replicare alla sua risposta, ma aggiungo: l'Italia è un eldorado in cui non c'è il proibizionismo? Sottosegretario Giovanardi, ma ha visto le carceri italiane?

Signora Presidente, con riferimento alla concessione demaniale marittima pluriennale intestata alla società Mondello Immobiliare italo-belga,

È tuttavia opportuno presentare un sintetico quadro esplicativo sul vigente riparto di competenze in materia di gestione del demanio marittimo nell'ambito della Regione Siciliana. L'entrata in vigore della legge n. 172 del 2003 ha sancito l'esercizio diretto delle funzioni gestorie delle aree demaniali marittime da parte della Regione, funzioni che, fino ad allora, erano state esercitate in regime di avvalimento dalle capitanerie di porto aventi sede nell'isola. Nell'immediatezza dell'entrata in vigore della citata stante la propria impossibilità di attendere alla gestione diretta dei beni del demanio marittimo, l'amministrazione regionale ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di poter autorizzare l'avvio

in scadenza al 31 dicembre 2010 (quindi alla fine di quest'anno), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato il menzionato supporto tecnico, escludendo qualunque attribuzione di responsabilità amministrativa in capo ai comandi periferici del Corpo, ricadente quindi esclusivamente sui competenti organi dell'amministrazione regionale. In merito ai contenuti dell'interrogazione, la capitaneria di porto di Palermo ha riferito che la società denominata Immobiliare italo-belga è titolare, in forza di atto pubblico n. 303 con scadenza 22 marzo 2012, di una concessione demaniale avente ad oggetto 36.000 metri quadri di suolo demaniale e 6.680 metri quadri di specchio acqueo situati in località Mondello del Comune di Palermo, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare. Con provvedimento n. 63 del 20 marzo 2009, emanato dall'assessorato regionale del territorio ed ambiente ai sensi dell'articolo 24 del regolamento al codice della navigazione, la citata società concessionaria è stata autorizzata a modificare l'assetto del suddetto stabilimento balneare attraverso la progressiva riduzione delle cabine balneari e una installazione di pedane in legno sulle quali collocare vari servizi (cabine, spogliatoi, bar, servizi igienici, La medesima società - previa comunicazione all'ente concedente - ha mantenuto, per l'intero anno, alla luce della facoltà di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2005, parte delle strutture in concessione sulle quali poter dare svolgimento ad attività collaterali alla balneazione. La Immobiliare italo-belga risulta, ad oggi, in regola con i pagamenti dei relativi canoni demaniali. All'interno dell'area in concessione insiste pertinenza demaniale marittima utilizzata dal concessionario quale sede del ristorante denominato Charleston, per la cui attività la concessionaria Immobiliare italo-belga ha stipulato un contratto di servizi con la società denominata Normanna scaduto il 31 dicembre 2009. Nonostante il mancato rinnovo del citato atto negoziale, la predetta Normanna ha continuato ad occupare i locali della ristorazione e contestualmente avviava un contenzioso in sede civile contro la Immobiliare italo-belga, rivendicando il proprio diritto possessorio sul bene demaniale in parola in ragione della pluriennale gestione dell'attività di ristorazione. Per contro, la Immobiliare italo-belga ha comunicato all'assessorato regionale territorio ed ambiente la cessazione del rapporto con la società Normanna e la indebita persistenza di personale della stessa nella struttura pertinenziale denominata Charleston. La Capitaneria di porto di Palermo, interessata dal predetto assessorato, ha acquisito gli atti del ricorso attivato dalla Normanna in base ai quali risulta come, sotto l'apparente forma del contratto di servizi, si celi in realtà un vero e proprio affidamento della gestione dell'attività di ristorazione, ascrivibile alla fattispecie di cui all'articolo 45-*bis* del codice della navigazione. In relazione agli sviluppi della tematica, come accertato dalla citata autorità marittima, la società concessionaria ha omesso di regolare la propria posizione con il ricorso all'autorizzazione di cui all'articolo 45-*bis* del codice della navigazione, incorrendo nella violazione dell'articolo 1164 del codice della navigazione, per la quale la capitaneria di porto ha elevato verbale di accertamento per la connessa fattispecie di illecito amministrativo. Nel contempo, tale infrazione è stata segnalata all'assessorato regionale territorio ed ambiente per l'eventuale avvio, nei confronti del concessionario, del procedimento amministrativo finalizzato alla decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 47 del codice della navigazione. Contestualmente, la Capitaneria di porto di Palermo, rilevando che la società Normanna permaneva *sine titulo*, con proprio personale, all'interno della struttura balneare, ha proposto all'assessorato territorio ed ambiente l'emanazione di un provvedimento ingiuntivo di sgombero nei confronti della menzionata società Normanna. Con nota del 16 marzo 2010, il citato organo regionale ha notificato l'ingiunzione di sgombero alla Normanna avviando, al contempo stessa data), nei confronti della concessionaria Immobiliare italo-belga la procedura per l'emanazione del provvedimento di decadenza, ai sensi dell'articolo 47 del codice della navigazione. In ragione di quanto argomentato si sottolinea, per quanto nelle dirette attribuzioni dell'autorità marittima e per gli aspetti che qui più rilevano, che l'azione della Capitaneria di porto di Palermo risulta essere stata circoscritta all'apprezzamento dei propri compiti di supporto tecnico prestato all'amministrazione regionale. In particolare, l'autorità marittima ha improntato il proprio ruolo alla scrupolosa osservanza del vigente dettato normativo, in stretta aderenza con gli indirizzi impartiti dal competente assessorato regionale, nel quadro delle misure di autotutela amministrativa ritenute opportune ed in linea con il rapporto di mero supporto tecnico alle attività di gestione che caratterizza, all'attualità, il riparto di competenze fra Stato e Regione sulla materia *de qua*, dal quale - si ribadisce - resta estranea qualunque attribuzione di responsabilità amministrativa ai comandi periferici del Corpo, permanendo quest'ultima in capo ai competenti organi della Regione Siciliana. Alla luce delle consolidate competenze regionali, infatti, si ritiene che l'apprezzamento dell'intera vicenda sia da ricondurre, in via esclusiva, alle valutazioni fatte dall'amministrazione regionale. Essa, nella fattispecie, assume, all'evidenza, il proprio fondamentale e legittimo ruolo di titolare delle funzioni gestorie degli ambiti demaniali marittimi, ciò fatte salve le iniziative discendenti dalle norme attributive delle competenze di polizia demaniale che l'autorità marittima continuerà, parallelamente, ad espletare, di pari passo con le attribuzioni che, sul piano del supporto tecnico-amministrativo, discendono dall'atto convenzionale che lega l'amministrazione regionale siciliana e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Proprio in virtù di tali competenze di polizia demaniale, in ogni caso, si assicura che l'autorità marittima continuerà a verificare la definizione dell'*iter* sanzionatorio proposto dalla stessa autorità marittima e avviato dall'organo regionale.

della quale mi ritengo soddisfatta. Prendo atto che l'amministrazione centrale ritiene che la responsabilità sia in capo alla Regione Siciliana, che è competente per materia. però, che la stessa non abbia preso in considerazione il fatto di migliorare l'utilità della gestione di un'area di ben 36.000 metri quadrati

per quelle città che hanno la fortuna di possederla, dovrebbe rappresentare - a mio avviso - il simbolo di una sana competizione tra più soggetti per offrire una migliore qualità del servizio, una diversificata fruizione dei luoghi; soprattutto dovrebbe essere uno spazio destinato non soltanto alla cittadinanza alla quale la spiaggia appartiene, ma anche al turismo che, con la sua industria, rappresenta un'immancabile occasione di crescita economica e sociale di tutta l'area.

significa creare un nuovo piano di utilizzo della spiaggia; significa mettere a bando le singole aree, creare nuovi lidi sul territorio e far nascere nuovi piccoli e giovani imprenditori, incrementando anche l'indice di occupazione e, soprattutto, creando un un modello competitivo per tutti i fruitori che si traduce poi, come sappiamo, in una migliore qualità del servizio. È evidente che tutto questo comporta anche nuovi introiti erariali per le casse regionali e la mancata adozione di provvedimenti in tal senso ha certamente mortificato ad oggi le casse della Regione con nuovi e possibili gettiti. Ricordo che già nel 1985 la capitaneria di porto aveva segnalato all'assessorato

Il 16 marzo di quest'anno, quindi dopo quasi 25 anni, sempre dopo segnalazione della capitaneria di porto, finalmente l'organo regionale si ravvede nei confronti della concessionaria Immobiliare italo-belga

Prendo atto con soddisfazione, ripeto ancora, degli accertamenti che gli organi preposti hanno effettuato, ribadendo la circostanza che la violazione in essere ha creato un *vulnus* da sanare con immediatezza per la corretta e legale fruizione di un bene così importante.

definizione dell'intero *iter* sanzionatorio proposto dalla stessa autorità marittima e avviato dall'organo regionale.

con riferimento all'atto ispettivo del senatore Di Giovan Paolo, inerente la situazione aziendale dell'agenzia GRT, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici dell'amministrazione che rappresento. La GRT - agenzia di stampa che fornisce contenuti giornalistici e servizi ad emittenti radiofoniche locali - risulta iscritta all'albo delle società cooperative ed è soggetta, in quanto tale, alla disciplina di cui alla legge n. 142 2001, recante revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. La stessa, in considerazione del servizio offerto, beneficia di sovvenzioni e finanziamenti pubblici. In particolare, la cooperativa gode, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di provvidenze all'editoria, di una riduzione al 50 per cento delle spese telefoniche sostenute per l'effettuazione della propria attività; la medesima, inoltre, beneficia dei contributi pubblici diretti alla stampa. Mi sembra importante, inoltre, fare presente che l'agenzia opera in stretto contatto con le emittenti radiofoniche locali, alle quali offre, previo abbonamento, informazioni giornalistiche. Fino allo scorso 27 febbraio (data a partire dalla quale detto contributo è stato soppresso) tali emittenti ricevevano dal Dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri l'erogazione di un contributo pari al 60 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei notiziari; in conseguenza di ciò, diverse emittenti radiofoniche hanno disdetto l'abbonamento sottoscritto con la GRT, che ha comunque manifestato la disponibilità a rivedere le condizioni contrattuali, con evidenti riflessi sul bilancio della medesima e, per ciò stesso, sulla possibilità di mantenere gli attuali livelli occupazionali. In proposito, informo che la GRT, per la realizzazione dei propri servizi, si avvale di un organico complessivo di 39 lavoratori tra soci, non soci e collaboratori esterni. Il competente ufficio del lavoro, sulla base dell'accesso ispettivo effettuato, ha reso noto che la società avrebbe compiuto, nel corso del 2009, due licenziamenti per giusta causa e per violazione dell'obbligo di esclusività delle prestazioni giornalistiche; dall'esame della documentazione acquisita nel corso degli accertamenti, emergerebbe anche che i rapporti tra l'agenzia e le organizzazioni sindacali non sono stati, in realtà, mai interrotti. In conclusione, nell'informare che, ad oggi, non risulta pervenuta presso l'Amministrazione che rappresento alcuna richiesta di valutazione della situazione aziendale all'attenzione, non posso che garantire la più ampia disponibilità a valutare, qualora richiesto, ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori.

che credo dia lustro anche alla nostra presenza qui, ricordando che domani, 16 aprile, ricorrono 22 anni dall'assassinio dell'amico e senatore Roberto Ruffilli, uno dei motivi per cui io sono qui ed è anche uno dei motivi per cui ho continuato a fare politica. Spero dunque che la Presidenza del Senato possa ricordarlo.

un collega bloccato per motivi di lavoro. Nell'analizzare la risposta, per la quale non esprimo né soddisfazione né insoddisfazione, perché siamo in una situazione di stallo, vorrei segnalare due cose. In primo luogo, che c'è un panorama giornalistico generale

la parte della cooperativa che è proprietaria anche di due radio esterne che sono tra i maggiori acquirenti dei servizi della cooperativa a livello giornalistico, ad un certo punto chiude i rubinetti dei contratti delle sue radio rispetto a quell'agenzia giornalistica

finestra"). Senatore Di Giovan Paolo, in merito alla sua richiesta riguardo al senatore Ruffilli, questa Presidenza informerà il Presidente e la Conferenza dei Capigruppo per le opportune decisioni.

nell'ambito delle iniziative assunte al fine di favorire la ripresa della vita accademica dell'Università degli studi de L'Aquila, la ricostruzione della Casa dello studente rappresenta per il Governo uno dei prioritari e significativi obiettivi per restituire alla città e soprattutto agli studenti dignità e speranza. Si ritiene, anche in questa occasione, di dover ancora una volta apprezzare l'operato della Protezione civile, del prefetto, delle istituzioni pubbliche locali e della Regione che si sono attivati per risolvere il problema dell'emergenza abitativa dei 14.124 studenti fuori sede iscritti nell'anno accademico 2008-2009, su un totale di 22.167. Come è noto al senatore interrogante lo stanziamento di 16 milioni di euro per la ricostruzione della Casa dello studente è previsto nel decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito dello stanziamento complessivo di 86 milioni di euro per gli edifici universitari danneggiati dal terremoto; la mancata erogazione dello stanziamento dipende dalle relative modalità indicate dall'articolo 14 del citato decreto legge, che prevede una complessa procedura che comporta anche una apposita delibera del CIPE. Riguardo al soggetto destinatario di tali fondi si fa presente che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto in parola, alla ricostruzione della Casa dello studente provvede il presidente della Regione Abruzzo, in qualità di commissario delegato, avvalendosi del competente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Questa priorità, è stato ricordato, dipende non solo dall'emotività che ruota intorno al problema della Casa dello studente - che è stata considerata un po' il simbolo della

che la Casa dello studente, ossia gli alloggi per gli studenti, deve avere nell'ambito della città universitaria dell'Aquila. Infatti, come ha ricordato lo stesso Governo, su oltre 22.000 iscritti all'università dell'Aquila,

il territorio - sono costretti al pendolarismo, in quanto le locazioni nella città dell'Aquila, per evidenti ragioni, sono impossibili o avvengono in un mercato della locazione che ha prezzi assolutamente inaccessibili per la gran parte degli studenti. signor Sottosegretario, era necessaria perché sia chiara l'importanza e soprattutto l'urgenza del problema. la mia soddisfazione è soltanto parziale, molto parziale, perché l'interrogazione verteva su tre aspetti importanti: l'aspetto dello stanziamento, quello dell'erogazione e quello della gestione dei fondi destinati e finalizzati alla realizzazione della Casa dello studente.

da circa un anno dal ministro Gelmini e dal presidente Berlusconi, fanno parte degli 86 milioni che nel decreto-legge n. 39 del 2009 sono finalizzati alle strutture universitarie.

per la ricostruzione della città dell'Aquila, ha previsto per l'erogazione di questi fondi una delibera adottata all'interno del Consiglio dei ministri, ed il Sottosegretario sostiene, a nome e per conto del Governo, che la costruzione della Casa dello studente è una priorità nel programma del Governo, non si riesce a comprendere per quale motivo

Per quanto riguarda poi la gestione dei fondi, ha fatto bene il rappresentante del Governo a ricordare che essa spetta al Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo,

ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 39 del 2009, per quanto riguarda le strutture pubbliche, in modo particolare quelle adibite all'istruzione e all'università. Ha poi ribadito la piena funzionalità del Presidente della Giunta regionale Abruzzo in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione dell'Aquila con l'ultimo decreto-legge, il n. 195 del dicembre scorso. Quindi, il mio vuole essere un invito al Governo

permette di rinnovare la memoria di quelle pagine di storia che interessarono i cittadini italiani dei territori dell'Istria, a ridosso dell'armistizio del 1943, ed è ormai inserito stabilmente nella programmazione scolastica, come può dedursi dallo spirito della nota indirizzata dal Ministero alle scuole lo scorso 2 febbraio e finalizzata all'attivazione di iniziative volte a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Le iniziative adottate dalle scuole coniugano, in genere, la ricostruzione, quanto più possibile accurata, delle vicende storiche con l'esigenza di ancorare a precise scadenze istituzionali concreti e non retorici elementi di educazione alla cittadinanza. Nel corso degli anni, queste iniziative vanno via via incrementandosi tant'è che nell'ottobre 2009,

da indirizzare alle istituzioni scolastiche, per una migliore conoscenza delle vicende che alla fine del secondo conflitto mondiale hanno riguardato il confine orientale italiano. Un primo impegno in tal senso si è concretizzato con il seminario nazionale «Le vicende del confine orientale ed il mondo della scuola» (seminario di formazione per studenti e docenti sulle tematiche collegate al Giorno del ricordo delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata), tenutosi in data 23 febbraio 2010 presso il Ministero, cui hanno partecipato numerose scuole di tutto il territorio nazionale e a cui ho personalmente presenziato, in rappresentanza del ministro Gelmini. Per l'approfondimento della storia degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, con nota del 4 dicembre 2009, sono stati segnalati alle scuole siti Internet di enti di studio e di ricerca che si occupano della materia. Compete comunque alle istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, avvalersi delle risorse professionali di istituzioni ed enti che abbiano sviluppato specifiche competenze in materia di ricerca storica e didattica, nonché dei testimoni diretti di tali tragici eventi. Faccio anche presente che la Commissione cultura della Camera dei deputati, con il parere favorevole del Governo da me espresso, il 18 febbraio scorso ha approvato una risoluzione con la quale impegna il Governo medesimo ad incrementare le iniziative nelle scuole su queste importanti vicende storiche. Ciò premesso, il Ministero, anche a seguito della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo in discussione, si è attivato presso tutti gli uffici scolastici regionali inviando il testo dell'interrogazione parlamentare e invitando gli uffici stessi a verificare ed eventualmente a segnalare se si siano verificati casi di mancata celebrazione del Giorno del ricordo, facendo conoscere gli eventuali provvedimenti adottati al riguardo. Alcuni uffici scolastici regionali (Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna, Umbria) hanno già comunicato che non risultano nel territorio di propria pertinenza casi in cui le istituzioni scolastiche hanno omesso di celebrare il «Giorno del ricordo»; al contrario, hanno fatto presente che gli istituti scolastici hanno dato vita ad iniziative di approfondimento sul significato dell'evento storico e sui fatti accaduti. Si attendono ora le comunicazioni da parte delle altre strutture periferiche. Da parte sua il rettore dell'Università degli studi di Roma ha fatto presente di aver effettuato verifiche presso le proprie competenti strutture, dalle quali non sono emerse circostanze quali quelle evidenziate dalla stampa. Il medesimo rettore ha anche precisato che laddove, come in casi analoghi alla ricorrenza del 10 febbraio siano prevedibili infiltrazioni di persone estranee alla comunità studentesca, l'Università adotta ogni opportuna misura atta a prevenire ed eventualmente contrastare possibili disordini. Quanto alla richiesta di istituire una commissione per effettuare una verifica dei libri di testo, vorrei far presente che la scelta dei testi scolastici avviene, di norma, attraverso una fase preliminare, nella quale si procede ad una verifica dei testi in uso, eventualmente anche nell'ambito di comitati misti docenti, genitori e studenti, in modo da valutare compiutamente le nuove proposte editoriali. Effettuata tale valutazione, i docenti interessati per materia, nell'esercizio della responsabilità connessa alla libertà di insegnamento, formulano le proposte che sono sottoposte, prima dell'adozione da parte del collegio dei docenti, all'esame dei consigli di classe, di cui fanno parte anche i genitori. Le regole vigenti assicurano, quindi, strumenti democratici di confronto e controllo, senza trascurare la circostanza che nell'attuale sistema scolastico, connotato dai princìpi propri dell'autonomia didattica ed organizzativa, non possono prevedersi interventi ministeriali in merito ai contenuti veicolati dai libri di testo, che rappresenterebbero un'interferenza impropria nella scelta degli autori da inserire nella programmazione didattica, scelta che deve essere invece operata dai singoli istituti. Compito del Ministero in materia di adozione dei libri di testo è soltanto quello di sostenere l'azione delle scuole con atti di indirizzo, rispettosi della sfera di questa autonomia che deve articolarsi ed estrinsecarsi - nelle diverse connotazioni, didattica, amministrativa, organizzativa e contabile - all'interno di un quadro di riferimento unitario al fine del perseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Anche quest'anno, con apposita circolare n. 23 del 4 marzo 2010, il Ministero ha fornito indicazioni in merito all'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2010-2011 richiamando i "vincoli" previsti per la loro adozione, quali la cadenza pluriennale, il rispetto dei tetti di spesa, la restrizione della scelta ai libri di testo a stampa per i quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, la progressiva transizione ai libri di testo *on line* e le scansioni temporali per le adozioni da parte dei collegi dei docenti.

da quanto riportato da alcuni importanti quotidiani della Capitale, che avevano riferito che il giorno 10 febbraio alcune classi scolastiche di importanti istituti si erano rifiutate

per anni ed anni la situazione di 350.000 nostri connazionali che dovettero lasciare quelle terre. Come ricordano anche la stampa e una serie

agli italiani che lasciavano quelle terre. L'impegno del Governo, del Ministero competente e in questo caso suo, gentile Sottosegretario, è quello del rispetto della legge:

di tutta la comunità italiana, che deve avere il coraggio delle sue azioni nei riguardi di propri conterranei e confratelli vilipesi, dimenticati ed offesi da un sistema che voleva nascondere quella situazione. Il signor Presidente della Repubblica lo ha segnalato in un incontro nel quale erano presenti personalità della cultura e dell'arte, che hanno onorato quelle terre e che hanno avuto dal Presidente della Repubblica un preciso impegno, che noi chiediamo al Governo di rispettare. Signor Sottosegretario, ringraziandola per il modo in cui ha dato

che lo riporti al livello del 2010. Inoltre, le chiedo di incrementare tale fondo per le difficoltà manifeste in cui si trovano le scuole. In particolare, bisogna mettere in campo un piano di rientro dei crediti che le scuole hanno nei confronti del Ministero della pubblica istruzione. In sostanza, il Ministero deve fare progressivamente fronte ai debiti maturati nei confronti delle autonomie scolastiche, che oggi ammontano a circa 1 miliardo di euro. Pertanto, come conseguenza, chiedo che venga modificato l'atto diramato alle scuole il 14 dicembre 2009, la nota n. 9537, relativa all'elaborazione dei bilanci delle scuole,

essendo state portate tutte le cattedre a 18 ore, non ci sono più insegnanti disponibili per quanto riguarda il completamento dell'orario laddove in una classe manchi ad esempio un insegnante. In quel caso, sa bene che le classi vengono scorporate, con grave danno per la didattica sia della classe stessa che delle classi in cui vengono immessi i ragazzi, con un danno rilevante per il funzionamento. Quei fondi attengono anche alle pulizie,

il minimo indispensabile per funzionare. Di questo stiamo parlando e lei sa bene che l'intero sistema scolastico pubblico viene tormentato, oserei dire umiliato, da questa mancanza costante di fondi anche per la sopravvivenza quotidiana. Lei sa cosa succede in tutte le scuole: vengono richiesti contributi ai genitori; tanti, troppi, anche a quelle famiglie che hanno difficoltà economiche; anche a quelle - pensi - che hanno l'esenzione dalla tassa scolastica. Eppure si chiedono contributi di 100, 200 euro perché manca tutto. Inoltre, quei contributi non sono più, come nel passato, da un lato volontari e dall'altro volti all'incremento della qualità scolastica, a quel di più che nel passato la scuola poteva permettersi (quale, ad esempio, il miglioramento dei laboratori, visite di istruzione particolarmente importanti, percorsi scuola-extrascuola): no,

hanno fatto fronte ai tagli con i contributi che avevano dato le famiglie e gli enti locali: avevano trovato un qualche rimedio a questa situazione in attesa di avere la restituzione di quello che invece non veniva restituito. Quando siamo andati al Governo abbiamo scoperto questa situazione, che potrebbe essere tecnicamente chiamata come debito fuori bilancio, cioè un debito di cui non c'era un resoconto nel bilancio dello Stato; abbiamo provato in due anni a farvi fronte riorganizzando la modalità di attribuzione delle risorse in due grandi capitoli, uno per il personale e l'altro per il funzionamento corrente, in modo da aumentare l'autonomia delle scuole, accorpando i capitoli di spesa ed evitando che, da un lato, si sommassero risorse non spese e, dall'altro, ci fossero invece importanti inadeguatezze e insufficienze di risorse. Tutto questo non è bastato. Avevamo aumentato le risorse insomma, la situazione stava iniziando ad essere ricomposta, un po' risistemata: rimaneva ancora un debito dell'ordine di 500 milioni di euro; ebbene, con il Governo attuale questo debito non è diminuito, non si è mantenuto il *trend* della diminuzione, ma è raddoppiato di 500 milioni di euro, che si aggiungono ai 500 precedenti. Le chiedo quindi di far fronte a questa situazione e le faccio delle proposte molto concrete, perché non voglio che tutto ciò si riduca ad una contrapposizione opposizione-maggioranza: avviamoci su delle proposte concrete. Non possiamo utilizzare l'autonomia scolastica come uno strumento su cui scaricare i debiti ed i tagli; l'autonomia scolastica non ha questa funzione.

pagando come Ministero ai Comuni ciò che devono avere per questa tariffa, questa tassa per i rifiuti solidi, ma anche di eliminare tutto ciò che non attiene alle autonomie scolastiche. Ad esempio, perché le scuole dell'autonomia debbono pagare i docenti gli esami di Stato, quando l'esame di Stato è una funzione propria dello Stato stesso che nulla ha a che vedere con l'autonomia scolastica? Facciamo sì che il fondo di funzionamento sia effettivamente legato allo svolgimento delle funzioni didattiche, delle innovazioni, alle esperienze innovative,

Dobbiamo avere rispetto, soprattutto per una grande istituzione nazionale come la scuola pubblica, che non può essere strozzata con queste modalità che la umiliano e le tolgono il futuro.

con la nota n. 9537 del 14 dicembre 2009 citata dall'onorevole senatore interrogante sono state fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche in merito alla compilazione dei documenti contabili per il programma annuale del 2010 tenendo conto delle risorse finanziarie alla data disponibili sui capitoli di spesa concernenti il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali. Ciò per consentire alle istituzioni scolastiche una programmazione certa con relativa copertura finanziaria. La nota in questione ha richiamato le istituzioni scolastiche ad una corretta tenuta delle scritture contabili mediante assunzioni degli impegni di spesa a tutela tutela dei beneficiari (personale scolastico, lavoratori socialmente utili, eccetera). Per quanto riguarda le supplenze è stata assicurata una risorsa complessiva annuale ad ogni istituzione scolastica, determinata sulla base dell'applicazione del decreto ministeriale n. 21 del 2007; le maggiori esigenze che saranno rappresentate dalle istituzioni scolastiche, previo controllo del fabbisogno segnalato, verranno soddisfatte in quanto deve essere assicurato il diritto all'istruzione. La circolare ha consigliato inoltre di applicare l'avanzo di amministrazione presunto nella misura necessaria e priva di vincoli al fine di consentire la copertura degli impegni assunti e da assumere dalla scuola. È stato segnalato a tale proposito che il bilancio dell'istituzione deve tendere al pareggio come previsto dal regolamento adottato con decreto interministeriale n. 44 del 2001. Per quanto concerne la rimodulazione dei contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie riguardante gli appalti storici (direttiva n. 68 del 2005), tale rimodulazione rappresenta il 2,25 per cento del totale delle risorse destinate a detti servizi; a tutte le istituzioni scolastiche sono assicurate risorse finanziarie quanto meno pari al costo del personale sostituito con i servizi esternalizzati, garantendo quindi i più opportuni livelli di servizio e liberando risorse per altre spese di funzionamento. Per quanto riguarda l'imputazione dei residui attivi nell'aggregato Z «Disponibilità da programmare», l'indicazione è data per i residui attivi vantati nei confronti del Ministero e per i quali sono state avanzate apposite richieste di assegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto concerne la copertura delle voci di spesa, i finanziamenti rientrano nell'assegnazione complessiva per spese di personale e di funzionamento; l'assegnazione dei fondi tiene conto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che gestiscono il *budget* assegnato sulla base dei criteri indicati nei decreti del Ministro. Vorrei anche far presente che in data 22 febbraio 2010 sono stati forniti ulteriori chiarimenti riguardo alle supplenze brevi e saltuarie, alla corretta assunzione degli impegni di spesa e alle spese di pulizia. A tale ultimo riguardo è stato confermato che a ciascuna istituzione scolastica viene garantita una risorsa finanziaria pari almeno al costo del personale statale ridotto per effetto della esternalizzazione dei servizi. Pertanto, nel caso in cui la somma per spese di pulizia, comunicata con nota del 14 dicembre 2009 protocollo n. 9537, fosse inferiore alla suddetta risorsa finanziaria, la stessa verrà integrata della differenza. Qualora dette somme già assegnate fossero eccedenti, rimarranno a disposizione della scuola per il prosieguo del contratto ex appalto storico, ovvero per le ulteriori esigenze di funzionamento. Infine, se la differenza tra le somme assegnate e il costo del personale ridotto per effetto della esternalizzazione stessa sia particolarmente rilevante, tale differenza sarà oggetto di opportuna analisi. In data 10 marzo scorso sono state anche fornite precisazioni ulteriori in merito alle richieste di maggiori finanziamenti per le spese di supplenze brevi che le istituzioni scolastiche debbono sostenere per consentire l'ordinato svolgimento delle lezioni e quindi garantire il diritto all'istruzione. È stato puntualizzato che la risorsa finanziaria già comunicata il 14 dicembre ultimo scorso comprende la spesa annua presunta per supplenze, determinata con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 21 del 2007. Dal decorso mese il Ministero procede periodicamente a monitorare gli impegni di spesa assunti nell'anno tramite i flussi finanziari al fine di eventuali reintegri. Il fabbisogno finanziario evidenziato verrà posto in rapporto alla spesa fissa che si sostiene in organico di diritto. Tale rapporto determina il tasso di sostituzione. Soltanto se il tasso di sostituzione è particolarmente elevato rispetto alle altre analoghe scuole,

Signora Presidente, non posso dire che il sottosegretario Pizza abbia colto le mie sollecitazioni. In particolare, mi dispiace che non abbia riconosciuto quali sono le reali difficoltà che stanno vivendo le scuole con questa carenza di risorse che le mette al di sotto

è un parametro che può essere utile per valutazioni di carattere generale, ma non può essere valido per attribuire le risorse, perché se in una scuola ci sono delle assenze realmente legate a motivazioni di salute o ad altro

per vedere se, effettivamente, esternalizzare le pulizie e la sorveglianza sia una modalità per far funzionare bene il servizio e, insieme, risparmiare risorse o se questo non sia assolutamente vero. Devo dire di aver vissuto molto male la polemica del Ministero sulla

la funzione del personale ATA è fondamentale nella scuola, sia per quanto riguarda la sorveglianza sia per quanto riguarda le azioni complessive di presenza rispetto ai ragazzi. Quindi, io sono molto d'accordo se andiamo a vedere gli effetti delle esternalizzazioni delle pulizie e